Il relatore facente funzioni, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

di autorizzare la ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti.

Noterete che questa ratifica arriva in maniera molto veloce.

di rafforzare la collaborazione con il Tribunale dei brevetti, garantendo l'immediata operatività sul territorio della nuova sede milanese. *(Brusìo)*. Mi fermo finché si placa il brusio.

e per la promozione della crescita delle imprese italiane nell'intero sistema Paese. L'accordo contenuto serve a consentire il corretto stabilimento ed il buon funzionamento

ed in prospettiva, poi, anche della sezione di Milano della divisione centrale. La divisione centrale viene creata a seguito dell'emendamento all'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti adottato dal comitato amministrativo il 26 giugno 2023,

un preambolo, che richiama l'Accordo del Tribunale unificato dei brevetti e il suo Statuto, disciplina le misure di sostegno che l'Italia deve fornire al Tribunale unificato dei brevetti sul territorio della Repubblica italiana precisa che l'obiettivo dell'Accordo stesso è di disciplinare le misure necessarie a garantire l'insediamento e il buon funzionamento degli uffici di Milano.

si parla di autorità italiane competenti, che sono ovviamente le autorità nazionali e locali dell'Italia, in accordo con leggi, regolamenti e disposizioni amministrative e consuetudini italiane; per "locali" si intende invece qualunque edificio o parte di esso che sia messo a disposizione del TUB; per proprietà del TUB, com'è evidente, si intendono tutte le proprietà, inclusi quindi non soltanto gli edifici di cui si parlava, ma i fondi, le entrate e altri beni, a qualunque titolo di possesso e in gestione; per familiari si intendono il coniuge o gli stretti familiari conviventi a carico del membro del personale TUB; infine, con il termine organizzazioni internazionali ci si riferisce alle organizzazioni aventi sede in Italia. L'articolo 2 disegna l'impegno italiano, che, come si diceva, consiste nel mettere a disposizione del TUB a titolo gratuito - questo va specificato - quale sede permanente della divisione i locali individuati dall'allegato 1 dell'Accordo. L'articolo 3 riconosce la personalità giuridica del TUB, come previsto dall'articolo 4 dell'Accordo, e in particolare la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili o immobili e stare eventualmente in giudizio.

i servizi di pubblica utilità necessari al suo funzionamento e abbia anche il più ampio accesso possibile alla rete Internet e a ogni altro canale di comunicazione. - ha il diritto di installare e gestire sistemi di telecomunicazioni nei locali. L'Italia si impegna a fornire le autorizzazioni necessarie a queste funzioni. Le spese di manutenzione dei locali destinati al TUB sono sempre a carico dello Stato italiano ed è facoltà delle parti stipulare eventuali intese supplementari per la migliore applicazione dell'Accordo e, in particolare, dell'articolo 4 di cui stiamo parlando. L'articolo 5 dispone l'inviolabilità dei locali e stabilisce dunque che nessuna pubblica autorità italiana possa avere accesso ai locali senza il consenso del Presidente della Corte di primo grado o persona da questo delegata. Tale consenso sarà presunto in caso di calamità naturali, incendio o altre situazioni emergenziali di questo tipo. L'articolo 6 stabilisce invece che le autorità italiane adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei locali (come, d'altra parte, è evidente ed ovvio). L'articolo 7 garantisce le comunicazioni, in particolare quelle dirette al TUB o al suo personale, e assicura a quelle ufficiali del TUB a quelle ufficiali del TUB i medesimi privilegi e le stesse immunità dei corrieri diplomatici (prima infatti abbiamo sottolineato anche l'inviolabilità della sede). L'articolo 8 riconosce al tribunale e alle sue proprietà, ovunque esse siano ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria. L'articolo 9 stabilisce la facoltà per il Tribunale di esporre la propria bandiera e il proprio emblema nei locali o sui mezzi di trasporto dallo stesso utilizzati in attività ufficiali, così come nei documenti di vario tipo o attraverso Internet e canali similari. L'articolo 10 si dedica invece alle agevolazioni finanziarie, in particolare il Tribunale unificato dei brevetti viene esentato, così come le sue proprietà, dalle imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, la nostra IVA, per acquisti di rilevante importo nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali. L'articolo 11 prevede esenzioni fiscali per un massimo di due veicoli acquistati o importati dal TUB per uso ufficiale ed ai relativi carburanti e lubrificanti. L'articolo 12 è relativo al personale e prevede, in particolare, il rilascio al personale stesso di una carta di identità che specifica lo *status* di titolare. L'articolo 13 prevede che, su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa autorizzare i familiari del personale del TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. Essi e i loro datori di lavoro sono soggetti, ovviamente, alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. È chiaro che le guarentigie, i privilegi, le immunità del TUB non si scaricano sui familiari che lavorino. Il regime previdenziale e sanitario del personale è regolato dall'articolo 14, mentre l'articolo 15 prevede che le autorità italiane facilitino l'ingresso ed eventualmente il soggiorno nel territorio nazionale dei membri del personale e dei loro familiari. 16 contiene una serie di disposizioni particolari, come per esempio l'obbligo di comunicazione alle autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, dell'elenco del personale e dei familiari reclutati L'articolo 17 dispone che per sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo sul TUB, l'Italia si impegna a fornire allo stesso il personale di supporto amministrativo per la divisione ubicata nel territorio del Paese e tale personale viene distaccato dalle amministrazioni pubbliche italiane secondo le leggi e i regolamenti italiani, e questo senza onere alcuno per il TUB. L'articolo 18 disciplina la responsabilità internazionale del Tribunale derivante dalle attività sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualunque atto o omissione da parte di rappresentanti, del personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni che è interamente in capo al TUB stesso e non sarà in carico all'Italia; quindi è una clausola di responsabilità. L'articolo 19 regola la risoluzione delle controversie sull'applicazione e interpretazione dell'Accordo, demandata a negoziati tra le parti e, se non vi è intesa, su richiesta di una o di entrambe le parti, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito all'uopo. L'articolo 20, infine, disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata. Le modifiche all'Allegato 1 entrano in vigore al momento della firma fra le parti.

oggi l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e recante la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo spazio economico europeo sottoscritto nell'aprile del 2014. Un Accordo che stabilisce gli opportuni adeguamenti affinché la Croazia sia inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo. Il disegno di legge di ratifica pone una clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

"Il link apre una nuova finestra") ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014***

intervengo soltanto per annunciare il nostro voto favorevole. Si tratta di un Accordo che va a completare la partecipazione della Croazia a tutti gli spazi dell'Unione e anche oltre. Devo soltanto annotare che la Croazia è stata molto rapida ad adeguarsi. Per esempio, pur essendo entrata nell'euro dopo di noi, ha già ratificato l'accordo MES, che purtroppo l'Italia ha mancato di ratificare, a a seguito delle decisioni di questa maggioranza. E ciò ha portato detrimento - io credo - alla nostra partecipazione all'Unione europea e alle decisioni che vengono prese di volta in volta, che ci trovano un po' come quello studente che viene messo con le orecchie da asino dietro la lavagna. Brava la Croazia che non l'ha fatto e, quindi, ratifichiamo questo Accordo e facciamo in modo che la Croazia partecipi a questo Spazio economico, che appartiene all'Unione e anche ai Paesi dell'EFTA.

la comunità europea a dare risposte positive anche agli altri Stati che fanno parte dei Balcani.

ritengo che ciò sia opportuno. Quindi rinnovo il voto favorevole a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle su entrambe le ratifiche. Signor Presidente, anche per noi l'Accordo non rappresenta né criticità, né oneri aggiuntivi. Pertanto, sinteticamente, annuncio il voto favorevole della Lega.

di un sempre maggiore coinvolgimento europeo, di un'Europa più aperta e inclusiva, efficace e democratica, unita, lo fa nella giusta maniera. Questo vale per la partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo, così come - me lo consentirà, Presidente per la coraggiosa, gridata voglia di Europa che hanno Paesi come la Georgia, con i cittadini che si riversano in piazza ogni sera a Tbilisi per resistere alla pressione russa per il cammino europeo di Paesi come la Moldavia, anch'essa nel mirino militare di Mosca, come i baltici e gli scandinavi; per la Bielorussia, schiacciata dal piede di Lukashenko ma non doma, in esilio o in prigione: a oggi, Presidente, sono 1.392 i prigionieri politici nelle segrete del regime;

duri, come il metallo della contraerea, a salvare vite umane. A Charkiv, a Odessa, a Chasiv Yar, a Kramators'k, a Druzhkivka, a Sloviansk, a Zaporizhzhia passa il confine dell'Europa, della sua anima, dei suoi valori di libertà e democrazia e della nostra dignità di democratici (di democratici, sì!), di parlamentari, di italiani, di cittadini europei, di esseri umani, di persone. Avete presente il concetto cristiano di persona? Ecco, la nostra dignità di persone passa di qui. Per questo, signora Presidente, per lo Spazio economico europeo che si gioverà del prezioso contributo della Croazia, così come per la Georgia libera, per la Moldavia, l'Ucraina combattente - l'Ucraina che resiste con loro fino alla fine, fino al ritiro completo dei russi dal suolo europeo di Ucraina *(Applausi) -* annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi)*.

voteremo a favore di questo Accordo illustrato minuziosamente dal collega Menia; un Accordo che ha a che fare con aspetti meramente pratici di una vicenda che però politicamente merita di essere sottolineata. L'arrivo a Milano del Tribunale dei brevetti, salutato da questo Governo con grandi squilli di tromba e di fanfare, è in realtà una grande sconfitta per il nostro Paese. Ricordiamo brevemente la storia: il Tribunale unificato dei brevetti e il brevetto unico europeo sono oggetto di una cooperazione rafforzata alla quale l'Italia e la Spagna non aderiscono nel 2013, al momento della creazione del brevetto unico e del Tribunale, perché è stabilito che, per poter registrare un prodotto con il brevetto unico, si debba fare in inglese, francese o tedesco. Quindi l'Italia - in modo secondo me sconsiderato - decide di restar fuori da questo meccanismo; fa anche una causa, insieme alla Spagna, davanti alla Corte di giustizia, che naturalmente perdiamo. Con il Governo Renzi - all'epoca il Sottosegretario competente era l'onorevole Gozi decidiamo invece fortunatamente di aderire a questo meccanismo, che è importante perché consente alle nostre imprese - non dimentichiamo di essere una delle più grandi potenze manifatturiere d'Europa - di poter tutelare la propria proprietà intellettuale con un meccanismo più semplice: si registra un brevetto in un Paese e lo si può difendere utilmente in tutti i Paesi dell'Unione europea. di una decisione logica, destinata a far bene soprattutto alle nostre imprese e, quindi, decidiamo di aderire. Ovviamente, essendo arrivati in ritardo, troviamo che la logistica di questo Tribunale era stata già ampiamente stabilita

Che cosa accade però? Come tutti ricordiamo, il Regno Unito esce dall'Unione europea ed evidentemente, uscendo da tutte le istituzioni europee, decide di rinunciare al Tribunale unificato dei brevetti. Milano, a questo punto, sarebbe stata la destinazione naturale per la nuova sede. Ricordo che l'Italia produce il 52 per cento dei farmaci di tutta Europa. Siamo una potenza manifatturiera sempre, ma nel chimico farmaceutico lo siamo assolutamente. Quindi cerchiamo di ottenere la sede di Londra, che semplicemente andava trasferita a Milano, così come è accaduto con l'Agenzia del farmaco, che da Londra dolorosamente andò ad Amsterdam per via del lancio della monetina. Vedo i colleghi del Governo di allora che ricordano ancora dolorosamente quel sorteggio. Invece Germania e Francia non hanno alcuna intenzione di mollare l'osso; quindi la trattativa va molto a rilento e si conclude con una soluzione di compromesso, che appunto il Governo illustra come un grande successo, ma che tale non è. Cosa accade? Di tutto il chimico farmaceutico che doveva andare a Londra, una parte, la chimica, viene unita alla meccanica e va a Monaco di Baviera. farmaceutica, invece, viene splittata in due parti e la parte cosiddetta assistita da SPC, che vuol dire *supplementary protection certificate*, che sono i farmaci che vanno sul bancone e venduti nelle farmacie, va a Parigi. A Milano arriverà soltanto il fitosanitario, l'alimentare e poco altro. Questa - secondo noi - è una decisione che certo porta qualcosa a Milano, ma che ancora ancora una volta dà un segnale. Ne parlavo prima, quando ricordavo che la Croazia è entrata nell'euro e ha ratificato il MES, mentre noi il MES non l'abbiamo ancora ratificato. Ciò dà proprio il segnale del nostro isolamento in Europa e del fatto che, quando ci si accompagna all'Ungheria, alla Repubblica Ceca o

nel margine. Certo siamo contenti. Io, figuriamoci, sono residente a Milano, sono milanese e sono ben contento che qualcosa arrivi e che l'edificio di via San Barnaba sia destinato al Tribunale unificato dei brevetti o a quello che ne rimane, con tutte le belle norme che il collega Menia ci ha indicato. Però non possiamo dimenticare che quello che doveva essere un passaggio molto semplice, cioè una sede del Tribunale

farmaci assistito da *supplementary protection certificate* non arriverà a Milano, ma andrà a Parigi, che aveva l'elettronica; bisogna trovare anche un nesso tra l'elettronica e i farmaci da bancone, ci vuole un certo impegno. Questa è la dimostrazione che si è mollato l'osso, pur di portare a casa qualcosa. Quindi, nel momento in cui ratifichiamo con soddisfazione l'accordo immobiliare, dobbiamo segnalare la disfatta sul piano dell'accordo politico.

È giusto - come hanno fatto i colleghi - ricordare un antefatto che riguarda il lavoro della Commissione politiche europee, quando io e il collega Scalfarotto abbiamo presentato una risoluzione, che poi è stata approvata all'unanimità dalla maggioranza e dall'opposizione, per dare più potere negoziale al Governo, recuperare un errore commesso in passato, quando, di fatto, il tema della sezione dei brevetti e marchi del TUB era stato attribuito a Monaco, a Londra e a Parigi, tagliando fuori l'Italia. Questa posizione ha dato più forza al Governo. Il fatto che a Milano vi sia una sezione distaccata è una buona notizia, ma non ci soddisfa del tutto perché avevamo chiesto che, oltre alla negoziazione della sede, ci fosse una rinegoziazione delle competenze. Ricordiamo che Milano non è solo la sede ideale per il tipo di attività che vengono svolte, ma anche per la parte industriale, per le nostre imprese. Si può avere un indotto di oltre 350 milioni di euro per quel territorio.

questa non è attinente puramente con la ratifica che - come è stato sottolineato - ha un valore pressoché amministrativo, consentendo al Tribunale di partire in maniera completa, è anche vero che era giusto capire in che modo si è arrivati sin qui e come sia necessario non fermarsi. È chiaro che siamo tutti contenti che Milano abbia ottenuto la sede. Siamo meno contenti che non siano state attribuite

che stiamo votando questa ratifica a fronte di una storia che il collega Scalfarotto ha riportato prima e che ci racconta di un Paese che ha scelto di non essere più di non appartenere più all'Unione europea, e che dimostra oggi invece come i Paesi che sono dentro l'Europa vogliono partecipare attivamente a quelle che sono regole comuni, rendendo tutti più forti e tutelando soprattutto i cittadini che appartengono a tali comunità e a un'Europa capace anche di tutelare. Questo lo dobbiamo dire. Pur votando favorevolmente e avendo l'orgoglio che sia Milano ad aver ottenuto questa sede, diciamo che è necessario un impegno in più. più. Milano si sta caratterizzando sempre di più anche con competenze molto specifiche rispetto a quelle che sono le scienze della vita. Sappiamo che lì c'è un polo grande e importante, che è quello che si è costituito anche nel dopo Expo, che sta dando grande valore alla Milano europea. Ed è per questo che noi chiediamo, pur votando favorevolmente al Governo, di insistere affinché quelle competenze che chiedevamo venissero assegnate a Milano, e quindi all'Italia, siano ribadite e chieste con maggior forza

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sento come un dovere etico prendere la parola per ricordare l'impegno civile e politico di un uomo Pio La Torre, che ha pagato con la sua vita la battaglia contro le mafie per la pace. Erano le ore 9,20 del 30 aprile 1982 e Pio La Torre si trovava in via Turba, a Palermo, insieme al compagno, amico e guardia del corpo Rosario Di Salvo, a qualche centinaio di metri dalla casa dov'era nato, nella borgata palermitana di Altarello. Fu aggredito da un commando mafioso mentre si stava recando alla sede del PCI regionale: morì all'istante sotto la raffica dei proiettili, mentre Rosario Di Salvo ebbe il tempo di estrarre la pistola e sparare cinque colpi, prima di perdere la vita. Deputato del PCI e sindacalista, dobbiamo all'impegno di Pio La Torre la costruzione di una nuova strategia di contrasto alle mafie che mirasse ad aggredire i patrimoni economici. È stato lui, infatti, il promotore di un disegno di legge che sarà approvato solo dopo la sua morte, che ha introdotto nell'ordinamento penale il reato di associazione mafiosa e previsti il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti, la legge che oggi conosciamo come Rognoni-La Torre. Non dobbiamo dimenticare che la lotta alla mafia per Pio La Torre fu anche difesa per la pace: la straordinaria mobilitazione contro l'installazione dei missili Cruise a Comiso nacque all'insegna di una richiesta di giustizia sociale e di una lotta contro tutti i poteri forti. Poche settimane prima dell'agguato, Pio La Torre era stato tra i promotori di una manifestazione per la pace e per il disarmo nucleare che vide un centinaio di migliaia di persone arrivare nella città siciliana. Tra le sue azioni, vi fu anche la firma di un'interrogazione parlamentare per chiedere conto dell'operato dell'operazione militare Trinacria 2. E difatti scoprì Gladio molti anni prima che venisse alla luce quel rapporto sommerso tra eversione nera, mafia, servizi segreti e massoneria. anni dopo il suo tragico omicidio, ricordiamo Pio La Torre perché il suo impegno politico, che ha spinto tanti di noi ad agire in prima persona nella società e in politica, rimanga vivo nella memoria e sia di ispirazione per le nuove generazioni: è grazie alla sua iniziativa politica che si è affermata la consapevolezza che la mafia non fosse solo una banda di delinquenti, ma anche una vera organizzazione criminale di una centrale economica sommersa. È grazie a lui se il reato di associazione mafiosa è entrato nel nostro codice penale. Come disse Enrico Berlinguer, subito dopo la sua morte, La Torre non era un uomo da limitarsi ai discorsi e alle analisi, ma faceva sul serio: per questo l'hanno ucciso. Oggi in quest'Aula ricordiamo Pio La Torre e, con lui, anche il suo amico e guardia del corpo Rosario Di Salvo, perché sono questi modelli, queste vite spezzate per combattere la comunità che devono disegnare la traiettoria del nostro impegno presente e futuro. Ai suoi funerali, dopo l'intervento commosso del presidente Pertini,

La lotta contro le mafie e l'impegno pacifista sono stati la sua grammatica civile e politica e sono l'eredità che dobbiamo coltivare ogni giorno.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, domani è il 1° maggio: dovrebbe essere la Festa del lavoro,

Tutti i giorni, in realtà, abbiamo notizie di questo tipo, anche se non sempre le cronache ce le restituiscono: spesso, magari, c'è un conto finale della giornata, ma continuiamo ad avere una

che stanno nel fatto che di prevenzione nei luoghi di lavoro ce n'è molto poca. Serve la formazione, ma non basta: bisogna prevenire, bisogna utilizzare risorse scelte che prevengano effettivamente quegli infortuni e - spiace dirlo forse bisognerebbe dedicare il tempo necessario a discuterne. Questa Assemblea, per esempio, i provvedimenti sulla sicurezza sul lavoro presenti nel decreto PNRR 2, non ha neanche avuto la possibilità di leggere e di discuterli; magari avremmo avuto delle proposte da fare

e dia risposte radicali. Ai morti non si può raccontare che forse un giorno vedremo e provvederemo, ma insomma va bene così. Bisogna dar loro risposte che diano certezza di prevenzione. ringrazio, senatrice Camusso, anche per aver richiamato la sicurezza sul lavoro come tema cruciale su cui questa Assemblea deve lavorare. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma il lavoro deve essere sicuro e la sicurezza deve essere garantita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

grazie.